Signor Presidente, onorevoli senatori, siamo assolutamente consapevoli della situazione di estrema difficoltà che sta attraversando il settore del florovivaismo ed è per questo che attribuiamo massima attenzione a una quota così significativa e strategica del comparto agricolo nazionale sia individuando ogni possibile strumento per un sostegno immediato sia lavorando in una logica di lungo periodo per il rilancio delle aziende del settore, compatibilmente con un'emergenza ed una crisi senza precedenti. Nelle continue interlocuzioni con le istituzioni europee, in particolare negli incontri bilaterali con il commissario all'agricoltura e in sede di Consiglio dei ministri, il Ministro ha sempre evidenziato la necessità di interventi urgenti ed efficaci a favore del florovivaismo. Per quanto concerne alcune prime misure introdotte, ricordo che nel cosiddetto decreto rilancio, oggi all'esame della Camera dei deputati, è previsto un contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, nonché l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 a favore delle imprese appartenenti alla filiera florovivaistica. Questi ultimi, inoltre, possono accedere alle garanzie offerte dal fondo Ismea, che ha una dotazione finanziaria finalizzata alle operazioni in periodo Covid di 350 milioni di euro. intenzione di questa amministrazione organizzare una campagna di comunicazione in Italia e all'estero per supportare il rilancio del prodotto florovivaistico *made in Italy*. Infine, per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole e della pesca che hanno subìto una forte crisi di liquidità, l'Ismea ha stanziato 30 milioni di euro per erogare prestiti di importo massimo pari a 30.000 euro a tasso zero e con durata di cinque anni, di cui i primi due di preammortamento. La misura va a sommarsi alle altre misure straordinarie assunte dall'Istituto, tra cui la sospensione delle rate dei mutui, l'estensione dell'operatività delle garanzie e l'allungamento dei termini per la partecipazione alla Banca della terra. La domanda potrà essere presentata tramite il portale dell'ISMEA direttamente dall'impresa interessata.

della cambiale agraria dell'Ismea che deve essere restituita? Ma non facciamo ridere, per non piangere, tutto il settore floricolo italiano!

al fine di sostenere le attività delle imprese del settore del florovivaismo, prevedendo l'istituzione di un fondo *ad hoc* (quello che voi avete negato nel decreto rilancio perché lo fate confluire nel Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi). A oggi non c'è una riga di contributo certo per il florovivaismo italiano. Sia chiaro che questo settore ha bisogno di un sostegno certo. Se voi non siete in grado di dare risposte agli italiani,

per i quali - a parere dell'interrogante - non è stata riconosciuta la possibilità di accedere alle misure di sostegno messe in campo dal Governo per sopperire all'emergenza Covid-19. Al riguardo, devo anzitutto sottolineare che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fin dall'inizio della pandemia, ha agito per assicurare la funzione degli strumenti di sostegno al reddito in favore di tutte le categorie dei lavoratori, al fine di contenere gli effetti catastrofici che la grave pandemia ha generato nel mondo del lavoro. Per tali ragioni, con il decreto-legge n. 18 del 2020 è stato introdotto un articolato sistema di tutele, che comprende tra l'altro l'erogazione d'indennità in favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti operanti in specifici settori produttivi. In particolare, l'articolo 29 prevede misure di sostegno in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. In merito all'interrogazione in oggetto, viene evidenziata la mancata erogazione delle indennità Covid-19 ai lavoratori con contratto a tempo determinato assunti nei settori del turismo e delle cure termali. Al riguardo posso riferire che l'INPS sta procedendo a un riesame e al conseguente accoglimento delle domande dei lavoratori, come sopra individuati, interpretando la disposizione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 e di cui al successivo articolo 84, comma 5, del decreto rilancio Italia, nel senso di ammettere al beneficio i lavoratori che oltre ad aver cessato involontariamente come stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020 - hanno avuto un ulteriore e ultimo rapporto di lavoro cessato involontariamente, ma non come stagionali e non necessariamente nei predetti settori produttivi. Voglio inoltre evidenziare che il Ministero del lavoro, d'intesa con il MEF, in questi giorni è impegnato nella predisposizione di misure atte a tutelare anche lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e delle cure termali, mediante l'emanazione di un decreto che dia attuazione all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 e che possa garantire una tutela

ha finalmente abbracciato questo tema, ma ritengo che bisognerebbe accelerare: qui si tratta di una platea non piccola, parliamo di almeno 180.000 persone che di fatto hanno lavorato nel settore turistico-ricettivo e termale nella precedente stagione, sono state assunte con contratto a tempo determinato e non stagionale - perché la norma consente all'imprenditore l'adozione di questo strumento - e sono senza protezione (quindi sono rimaste scoperte per i mesi di marzo, aprile e maggio). Credo abbiamo la necessità di accelerare: ho parlato già qualche altra volta con il Ministro che ha accennato a quest'intervento normativo, ma ravviso la necessità di spingere, perché non possiamo lasciare ancora senza alcun sostegno una platea tanto vasta, giacché peraltro la stagione turistica incerta, ormai avviata, probabilmente non consentirà l'assorbimento di tutte queste persone, che si ritroveranno in autunno a non poter nemmeno dimostrare la stagionalità del rapporto di lavoro.

Presidente, nell'ambito delle strategie di prevenzione, assistenza e controllo del contagio da coronavirus, l'Istituto superiore di sanità ha promosso la *survey* nazionale sul contagio nelle strutture residenziali e sociosanitarie. Nella Regione Lombardia sono state contattate

3.045 residenti, dei quali 166 Covid-19 positivi e 1.459 con sintomi compatibili. Più in generale, nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS-Cov-2, fin da subito è emersa la necessità di prestare massima attenzione nei confronti della popolazione anziana. Sin dall'adozione del decreto del anche per la Regione Lombardia è stata prescritta la rigorosa limitazione all'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali quale fondamentale misura di prevenzione del contagio. Le persone anziane rappresentano la popolazione più fragile per eccellenza da proteggere con le più idonee cautele, anche e soprattutto nel corso dell'epidemia che stiamo vivendo. La circolare del Ministero della salute del 25 marzo 2020, recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza Covid-19», ha segnalato l'emergenza connessa agli ospiti e i pazienti ricoverati nelle RSA, soggetti particolarmente fragili per i quali è necessario effettuare una stretta sorveglianza, nonché il rafforzamento dei *setting* assistenziali. La circolare ha posto in rilievo le seguenti e indispensabili azioni: azioni: prioritariamente le strutture residenziali dedicate ove trasferire i pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; potenziare il personale in servizio presso queste strutture, anche attraverso meccanismi di reclutamento straordinario, nonché la possibilità di ricorrere a personale già impiegato nei servizi semiresidenziali e domiciliari, predisponendo percorsi formativi e di prevenzione specifica per tutto il personale ivi operante; effettuare sistematicamente tamponi per la diagnosi precoce dell'infezione a carico degli operatori sanitari e socio-sanitari e dotarli di dispositivi personali di protezione. Occorre, inoltre, garantire la continuità dei servizi di mensa, lavanderia, pulizia e servizi connessi, estendendo anche agli operatori dedicati le misure mirate a definire un'eventuale infezione. La successiva circolare ministeriale del 29 marzo 2020, recante «Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-Cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie

e ai rischi di esposizione professionali, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico del Covid-19. Allo scopo di perseguire l'obiettivo volto alla massima tutela possibile, è necessario che il personale sia dotato, in base alle evidenze scientifiche, di dispositivi di protezione individuale di livello adeguato al rischio professionale a cui viene esposto e ciò, maggior ragione, per quanto concerne il personale chiamato a operare in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio. Sul versante dell'effettuazione dei test, la circolare n. 11715 del 3 aprile 2020, recante «Pandemia di Covid-19 - aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità», ha raccomandato che l'esecuzione del test venga assicurata agli operatori sanitari e assimilati a maggior rischio sulla base di una definizione operata dalle aziende sanitarie quali datori di lavoro. Inoltre, tra gli operatori esposti a maggior rischio cui effettuare effettuare il test per tutelare loro stessi e per ridurre il rischio di trasmissione nosocomiale, sono stati individuati anche quelli delle RSA e delle altre strutture residenziali per anziani sebbene asintomatici. Desidero segnalare che il documento dell'Istituto superiore di sanità «Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie», aggiornato al 17 aprile 2020, è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome con la circolare del Ministero della salute del 18 aprile 2020. Le indicazioni del documento riguardano gli ambiti della prevenzione e preparazione delle strutture residenziali alla gestione di eventuali casi sospetti, probabili o confermati. Le misure prevedono un rafforzamento dei programmi e dei princìpi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, inclusa un'adeguata formazione degli operatori. In particolare, il rafforzamento deve prevedere un'adeguata preparazione della struttura per prevenire l'ingresso di casi Covid-19 e per gestire eventuali casi sospetti, probabili o confermati che si dovessero verificare tra i residenti. Il documento contempla la necessità di un'adeguata sorveglianza attiva tra i residenti e gli operatori per l'identificazione precoce di casi. Le strutture devono essere in grado di effettuare un isolamento temporaneo dei casi sospetti e, in caso di impossibilità di un efficace isolamento per la gestione clinica del caso confermato, di effettuare il trasferimento in ambiente ospedaliero o in una struttura adeguata all'isolamento per ogni ulteriore valutazione clinica e per le cure necessarie. Per quanto riguarda gli aspetti di rilievo regionale, l'assessorato al *welfare* e la direzione generale *welfare* della Regione Lombardia hanno segnalato quanto segue. La gravissima pandemia ha colpito in modo particolarmente particolarmente severo la Regione, che ha una percentuale di popolazione anziana tra le più alte in Italia, con gli *over* 65 pari al 22,5 per cento della popolazione, in base alla fonte Istat del 1° gennaio 2019. Le RSA destinate ad accogliere quasi esclusivamente cittadini ultrasessantacinquenni al 31 dicembre 2019 erano 708, di cui 657 gestite da privati, per un totale di 64.411 posti letto. Per fronteggiare l'emergenza sanitaria, la Regione riferisce di aver tempestivamente fornito una serie di istruzioni operative impartite alle varie articolazioni del servizio sanitario regionale ed aggiornate costantemente per recepire le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali. La Regione precisa di aver adottato le procedure per l'effettuazione dei tamponi agli operatori e ai pazienti ospiti in linea con le disposizioni ministeriali e di avere costantemente fornito indicazioni aggiornate al personale sanitario circa le varie misure di prevenzione e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. familiari degli ospiti nelle RSA, la Regione ha disposto le prime misure di limitazione alle visite con la comunicazione diramata il 23 febbraio 2020, dove si precisa che i parenti dei pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie e sociosanitarie devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad uno per paziente. La Regione Lombardia esclude, inoltre, di avere adottato misure tali da favorire indebite commistioni nella gestione di pazienti Covid positivi o sospetti Covid con quelli negativi, e riferisce di avere consigliato alle strutture il blocco dei nuovi accessi dal 9 marzo 2020 e l'individuazione di strutture autonome dal punto di vista strutturale (padiglione separato o struttura fisicamente indipendente) ed organizzativo, al fine di assicurare assistenza a bassa intensità ai pazienti Covid-positivi. L'adesione è stata comunque su libera scelta degli enti. Specifiche misure di tutela, prevenzione e cura degli ospiti delle RSA e di sicurezza per gli operatori coinvolti sono state previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. XI/3018 del 30 marzo 2020, la quale ha auspicato, in particolare, che a beneficio degli ospiti particolarmente particolarmente fragili accolti nelle RSA le cure fossero prestate presso la stessa struttura, onde evitare i rischi dovuti al trasporto esterno. Inoltre, la Regione Lombardia, con il decreto n. 529 dell'11 aprile 2020, a firma del presidente regionale, ha costituito una commissione di verifica per le RSA composta da eminenti personalità scientifiche esterne alla Regione. Essa ha il compito di effettuare un *audit* strutturato, al fine di verificare le migliori *best practice* e le azioni eventualmente necessarie per affrontare al meglio nel prossimo futuro una convivenza con il virus Covid-19. ha dato mandato alla *task force*, costituita in seno all'unità di crisi, di procedere ad effettuare accurate verifiche ispettive presso le RSA di diverse Regioni. Allo stato attuale, tali verifiche sono state avviate in Lombardia, Calabria e Sicilia, in riferimento a specifiche situazioni di contagio o decesso verificatesi in alcune strutture In particolare per quanto riguarda la Regione Lombardia, in data 9 aprile 2020, ha avuto luogo una visita ispettiva del Ministero della salute presso il Pio Albergo Trivulzio, all'esito della quale sono state riscontrate criticità di tipo organizzativo e gestionale. In data 20 maggio 2020, il Ministero della salute ha inviato alla Regione Lombardia una nota contenente le prescrizioni relative alle azioni di miglioramento da implementare per superare le criticità emerse, volte in particolare alla tutela dei soggetti fragili che rappresentano l'elemento più debole e quindi più a rischio nella catena del contagio. È stata inoltre segnalata la necessità che la Regione Lombardia si adoperi per attivare ed implementare tutte le azioni previste e dettate dalla circolare del Ministero della salute del 17 marzo 2020, e successive integrazioni, come pure dal documento elaborato dall'Istituto superiore di sanità, aggiornato al 16 marzo 2020, parimenti richiamato. La Regione Lombardia è stata altresì invitata a comunicare i tempi di adeguamento alle predette prescrizioni. Assicuro che è preciso intendimento del Ministero della salute effettuare ulteriori attività di verifica presso tali tipologie di strutture assistenziali territoriali, al fine di fare luce sulle criticità organizzativo-strutturali e di sicurezza che abbiano potuto concorrere al diffondersi del contagio tra i degenti e tra questi e gli operatori sanitari, nonché di verificare, nel contempo, se le misure adottate da parte delle Regioni in materia di RSA siano state e siano aderenti a quanto dettato dalle specifiche circolari emanate dal Ministero della salute. Da ultimo, rilevo che con l'inizio delle fasi successive al *lockdown*, in cui comunque vi è la convivenza con il virus ed un graduale ritorno alle normali attività, diventa indispensabile un rimodellamento dell'assistenza che consenta un tempestivo intervento in caso di nuovi focolai, con una presa in carico dei pazienti affetti e di quelli in isolamento domiciliare, anche attraverso una reale integrazione tra assistenza ospedaliera ed assistenza sul territorio. Inoltre, è necessario garantire la continuità assistenziale per i pazienti fragili (cronici, non autosufficienti e disabili), assicurando il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute dei pazienti e degli operatori attraverso eventuali specifici protocolli. Tali priorità hanno costituito l'oggetto di un recente intervento normativo di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 34 del Va anche ricordato che presso il comitato tecnico-scientifico è attivo un tavolo di lavoro che sta sviluppando linee guida che rendano omogenee in tutto il territorio nazionale le iniziative regionali in tema di rafforzamento dell'assistenza territoriale e la sua integrazione con quella ospedaliera, tenendo conto delle specifiche esigenze sopra ricordate. Rassicuro pertanto i senatori interroganti che massima è l'attenzione riservata dal Ministero della salute circa il rispetto delle migliori pratiche di gestione delle RSA nel presente contesto emergenziale. Per concludere, chiedo scusa al senatore Mirabelli perché i dati che mi sono stati forniti dal Ministero sono aggiornati al 14 aprile 2020. Ho già sollecitato tempo fa dati aggiornati. Credo che avere dati aggiornati possa essere utile per capire se dal 14 febbraio ad oggi le cose sono notevolmente migliorate o no, quindi sarà mia premura, appena i dati saranno in nostro possesso - quindi trasmessi dalle Regioni e analizzati - fornirli per un'accurata analisi. *(Applausi)*.

Governo per aver ribadito la volontà di tenere aperto un *focus* sulla vicenda delle case di riposo in generale dopo quello che è successo con la pandemia. che presenteremo un'altra interrogazione per avere dati più aggiornati rispetto alla situazione delle case di riposo. Prendo atto anche delle risposte pervenute dalla Regione Lombardia che lei ci ha riferito (credo che i dati le venissero, appunto, dalla Regione). Ne prendo atto e registro che continuano essere autoassolutori.

nelle case di riposo, la percentuale di mortalità è stata del 9,7 per cento per malattie legate al Covid, mentre nel resto d'Italia è stata del 3,7 per cento. Qualcosa non ha funzionato noi dobbiamo capire che cosa non ha funzionato, ripeto, non per attribuire le responsabilità a qualcuno - a questo ci pensa la magistratura - ma perché vanno corretti quei meccanismi che non hanno funzionato e perché, se l'epidemia riparte, dobbiamo essere sicuri che quegli errori non verranno rifatti. Lo dobbiamo ai cittadini lombardi e ai cittadini italiani. Se non facciamo questo e ci limitiamo - come purtroppo ho sentito dalle risposte che ci ha riferito - ad autoassolverci e a dire che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo che dovevamo fare, quel dato del 9 per cento - rispetto al 3 per cento nel resto d'Italia - continua a non spiegarsi e siccome non penso che la sfortuna sia una categoria di cui possiamo appropriarci,

alle quali risponderanno il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'istruzione. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Con il decreto ministeriale 23 dicembre 2015 recante regole tecniche di attuazione della CIE sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta di identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato. Nella Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe partire a breve il servizio di emissione da parte dei Comuni della nuova CIE in forma trilingue: italiano, inglese e tedesco. L'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, prevede che: «Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonché per le frazioni Oltretorrente,

che saranno rilasciate dai Comuni citati in quanto le dotazioni *software* fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato non la prevedono. Si chiede, quindi, di sapere quali siano i motivi per i quali nell'emissione delle nuove carte d'identità elettroniche non si sia tenuto non si sia tenuto conto delle specificità linguistiche presenti in Trentino-Alto Adige-Südtirol come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, citato e se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere in tal senso.

senatore interrogante richiama l'attenzione sul servizio di emissione della nuova carta d'identità elettronica avviato nella Provincia autonoma di Bolzano, ponendo l'accento sulla previsione normativa contenuta nel decreto del che prevede che la stessa venga emessa in alcuni territori comunali in lingua italiana, tedesca e ladina, oltre che in inglese, lingua predefinita dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2015. Nel mese di maggio è stato avviato presso il Comune di Bolzano il rilascio della carta d'identità elettronica bilingue italo-tedesca. Ciò è il frutto di un percorso che ha coinvolto il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e il Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige. È particolarmente complesso sotto il profilo tecnico amministrativo, in quanto ha comportato la necessità di adottare l'impostazione grafica e gli *standard* tecnici definiti per la carta d'identità elettronica a livello nazionale in modo da corrispondere al peculiare assetto autonomistico presente in quei territori. Il documento d'identità ha assunto la veste grafica plurilingue e tale caratteristica ha necessariamente comportato difficoltà nell'elaborazione dello schema dei testi e delle formulazioni da riprodurre in modo da comprendere caratteri grafici identici e l'utilizzo di una terminologia che è stata condivisa con i rappresentanti istituzionali dei diversi gruppi linguistici interessati. A seguito della positiva conclusione della realizzazione della carta d'identità elettronica italo-tedesca, si può ora procedere ad approfondire la progettualità della carta d'identità con traduzione in lingua ladina, ivi compreso il formato della stessa. A tal fine potrà rendersi necessaria una modifica tecnica al citato decreto ministeriale del 2015 per una specifica configurazione del supporto per la carta italo-tedesco-ladina perché lo stesso dovrà essere predisposto per l'introduzione di quattro, lingue italiano, inglese, lingua predefinita, tedesco e ladino, nel rispetto della previsione dell'articolo 32 decreto del Darò quindi un personale impulso ai necessari ulteriori approfondimenti al fine di consentire anche il rilascio della carta d'identità con la lingua ladina. Ritengo comunque di segnalare che nelle more della definizione dei necessari aspetti aspetti tecnici propedeutici all'avvio delle attività di emissione del documento, il commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, unitamente al consorzio dei Comuni, ha già predisposto in lingua ladina le note di trasmissione e le istruzioni di attivazione della carta d'identità elettronica bilingue italo-tedesca, al fine di agevolare i cittadini residenti nei territori della Val Gardena e della Val Badia nell'utilizzo del documento. Quanto sopra nel doveroso rispetto della normativa vigente che si ispira al riconoscimento e alla tutela delle minoranze linguistiche quale principio fondamentale della nostra Carta costituzionale.

anche in lingua ladina nei Comuni dove è insediata la rispettiva minoranza linguistica. L'auspicio - che ho visto è comune - è di poter risolvere in termini brevi i problemi tecnici cui ha fatto cenno, considerato che si tratta comunque di valori protetti

anzitutto il Ministro per la sua presenza. Nella mia interrogazione sottopongo alla sua attenzione la questione del rilascio della carta d'identità per i bambini delle cosiddette famiglie arcobaleno. In data 3 aprile 2019 veniva pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* una direttiva dell'allora Ministro dell'interno che modificava le disposizioni di un altro decreto ministeriale del 2015 e ripristinava la dicitura «padre e madre» sui documenti d'identità dei minori, con particolare riferimento alle carte elettroniche necessarie

presentate congiuntamente da padre e madre allo sportello anagrafico. Accadde così che nel 2019 venivano immediatamente adeguati tutti i testi della modulistica e anche del sistema elettronico, con la conseguenza che soltanto le domande supportate da due genitori di sesso diverso venivano accolte e sono tutt'oggi accolte. È noto a tutti, non solo in quest'Aula, che la presenza di due genitori di sesso diverso non è una condizione comunque presente nella vita di tutti i minori. Penso semplicemente, senza voler andare troppo lontano, ai minori orfani. In particolare, esistono nel nostro ordinamento bambine e bambini che, per effetto di iscrizioni anagrafiche o in casi particolari di sentenze di adozione già passate in giudicato

due genitori dello stesso sesso, i quali si trovano oggi nell'impossibilità di richiedere e ottenere per i loro figli un documento di identità corrispondente all'identità personale e sociale; nell'imminenza Come sapete, il testo è depositato e io chiedo di sapere dal ministro Lamorgese semplicemente se si può ripristinare la dicitura esistente prima del 2019, quando le parole: «padre e madre» erano semplicemente indicate con la parola: «genitori».

richiama l'attenzione su alcune criticità che sarebbero derivate dalle modifiche apportate in materia dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019. Con il predetto provvedimento sono state adottate modifiche al precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2015, che hanno ripristinato sulle carte d'identità elettroniche dei minori valide per l'espatrio le diciture: «padre e madre» in luogo della dicitura: «genitori». Gli elementi riportati sulla carta d'identità rappresentano i dati anagrafici del titolare risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza e conforme ai rispettivi dati dello stato civile, nonché ai relativi registri. Evidenzio che il 9 gennaio scorso il TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione di quattro ricorsi giurisdizionali volti ad ottenere l'annullamento delle disposizioni del decreto ministeriale del 2019, ritenuto illegittimo per violazione di plurime disposizioni di legge. Ad oggi non risulta che i ricorrenti abbiano riassunto le cause dinanzi al competente giudice ordinario. Il Garante per la protezione dei dati personali ha di recente comunicato di aver ricevuto segnalazioni in merito a delle criticità nell'applicazione del decreto ministeriale del 2019, in relazione ai profili riconducibili alla protezione dei dati e alla tutela dei minori, manifestando la disponibilità per l'individuazione di interventi finalizzati alla loro soluzione. abbiamo accolto la disponibilità dell'Ufficio del garante per un approfondimento della tematica e informo che già nei prossimi giorni sarà avviato dai competenti uffici del Ministero un confronto sul tema. All'esito delle interlocuzioni potranno essere definiti gli ambiti di intervento che dovessero evidenziarsi necessari. Una volta pervenuti a una complessiva valutazione sul tema, potrà essere considerato il conseguente adeguamento dei *software* idonei a immettere i dati relativi alle domande di rilascio della carta d'identità elettronica per l'espatrio da parte di coppie omogenitoriali, essendo comunque necessaria una previa modifica regolamentare.

dell'ideologia che un Governo ritiene di portare avanti rispetto ad uno precedente, esistono dei diritti inviolabili che in questo momento vanno rispettati in riferimento a questi bambini che sono ancora di serie B, in un Paese nel quale basta avere la fortuna di nascere da una coppia eterosessuale per accedere a tutti i diritti. Questi bambini non hanno i nonni, né gli affini, vengono puniti per il modo in cui sono nati e per l'amore dei loro genitori. Credo che che in un Paese laico, libero e democratico ciò non possa continuare ad accadere.

Lei, signor Ministro, sulla condanna a Silvio Berlusconi nel processo sui diritti TV Mediaset e sulle dichiarazioni del giudice Amedeo Franco ha scelto la linea del silenzio: non ha proferito alcuna parola. Noi non le contestiamo questo, figuriamoci; le abbiamo contestato in passato l'opposto, cioè l'eccessiva loquacità, per un Dicastero che necessiterebbe di maggiore sobrietà. Il problema non è infatti che non abbia detto nulla, ma semmai che non abbia fatto nulla. Il *question time* di oggi è uno strumento che utilizziamo per sollecitarla a fare. Il giudice che si sfoga, che parla di porcheria, di plotone di esecuzione e di sentenza *a priori* è l'estensore della sentenza che ha condannato il presidente Berlusconi, con evidenti ricadute nel gioco democratico del Paese, perché quella sentenza ha tenuto fuori dal Parlamento l'uomo che ha guidato più a lungo un Governo nella storia d'Italia, e lei non può fischiettare e girarsi dall'altra parte, come se nulla fosse accaduto. Non tocca a noi dire come sono andate le cose, ma tocca a lei dare un contributo decisivo per scoprire la verità. Non ci appassionano le tifoserie, ma nemmeno l'omertà che rende tifosi al contrario. Non possiamo permetterci di minimizzare e non possiamo accettare che questa storia finisca nei trafiletti dei giornali, quando in passato è stata stampata nelle prime pagine di tutti i quotidiani. La sentenza Berlusconi è la cartina al tornasole del funzionamento della giustizia italiana, per un ex Capo di Governo così come per un cittadino qualunque. Noi dobbiamo avere la certezza dell'imparzialità della giustizia nel nostro Paese; ne va della credibilità e dell'autorevolezza della magistratura, già duramente colpita. E tutte le forze politiche dovrebbero pretendere trasversalmente, anziché il brusio, anche un po' fastidioso, alla mia sinistra. Do un valore in più al fatto che a sollecitarla in questo senso non sia solo il partito di Berlusconi, ma un partito diverso, che mette al centro il garantismo e il rispetto dei cittadini davanti alla legge. Quindi, signor Ministro, le chiediamo che azioni intende intraprendere concretamente per accertare come sono andati realmente i fatti. Signor Presidente, gli interroganti fanno riferimento a una registrazione diffusa da organi di stampa e attribuita al magistrato dottor Amedeo Franco, deceduto nel maggio 2019, per chiedere quali iniziative il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda adottare al riguardo. Mi soffermo proprio sulle attribuzioni del Ministero per ricordare che, in generale, secondo il decreto legislativo n. 109 del 2006 il Ministero della giustizia compie accertamenti tendenti a chiedere eventualmente l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del competente organo istituzionale a ciò preposto davanti al Consiglio superiore della magistratura, cioè la procura generale presso la Corte di cassazione. L'accertamento deve muovere da fatti circostanziati e specifici, relativi esclusivamente a magistrati attualmente in servizio. Con riferimento alla vicenda oggetto di interrogazione, laddove dovessero emergere profili fattuali di questo tipo, nella cornice di competenze e nel quadro normativo che ho appena evidenziato, gli uffici effettueranno tutte le valutazioni del caso nel termine annuale loro assegnato. *(Applausi)*.

credo che il suo atteggiamento in altre circostanze sia stato ben diverso, anche in fattispecie che sono molto simili da quella di cui stiamo discutendo oggi. Devo dire che non mi convinceva l'idea di una Commissione parlamentare rispetto a questo tema, perché credevo che all'interno del Dicastero e nelle azioni del Ministero della giustizia si potessero già espletare tutte le attività necessarie per cercare di fare chiarezza su una vicenda che è abbastanza pesante per il nostro Paese, al di là di come finirà questa storia. Non è detto che ci sia una via soltanto rispetto a quello che viene che viene discusso rispetto a questo tema, ma sicuramente l'accertamento della verità è una necessità che avvertiamo tutti. Se il Ministero della giustizia decide di non fare nulla

*(FIBP-UDC)*. Signor Ministro, ben comprendo i suoi impegni e la sua responsabilità in un settore così delicato e vitale per il funzionamento dello Stato e della democrazia (vedi interrogazione precedente). Le chiedo però di andare oltre la relazione predisposta dai suoi uffici e senz'altro da lei visionata in risposta alla mia interrogazione. Le normative anti-Covid (decreti-legge, DPCM, ordinanze e decreti) mirano ad evitare assembramenti e a praticare il distanziamento sociale. I tribunali soffrono cronicamente di mancanza di spazi. Nel contratto di Governo del Conte 1 era prevista la revisione dei tribunali soppressi; il decreto legislativo n. 155 del 2012, articolo 8, comma 4-*bis*, prevede che il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie. Allora la riforma del 2012 si può rivedere e dare inizio alla procedura di riapertura dei trenta tribunali soppressi su e giù per l'Italia, utilizzando intanto gli immobili, come uffici giudiziari periferici e sedi distaccate dei tribunali accorpanti, al fine di garantire il funzionamento della giustizia. Emblematico è il caso della Provincia di Cuneo, dove su quattro tribunali tre sono due a Mondovì e Saluzzo accorpati a Cuneo ed Alba accorpato ad Asti. Il fabbricato di Alba, pressoché nuovo e funzionale, è a disposizione, previo accordi con la Regione e con il Comune, essendo al centro di area economicamente forte e con un bacino di 200.000 abitanti, essendo la vecchia giurisdizione del tribunale di Alba estesa anche a una parte della Provincia di Torino. È prevedibile che la prevenzione antipandemia non sia breve. Sperando che la fase acuta sia passata in tutto il mondo e la malattia sia in remissione, andiamo però senz'altro verso un nuovo stile di vita e nuove abitudini nei rapporti sociali.

soppressi su e giù per l'Italia, non comprendendo ancora oggi le ragioni della riforma né sotto l'aspetto economico, né sotto l'aspetto funzionale. Attendo pertanto fiducioso una sua risposta e la ringrazio.

che si intendono intraprendere per assicurare che nell'ordinario svolgimento dell'attività giudiziaria vengano rispettati i protocolli di prevenzione per il Covid-19, essendo stati anticipati al 30 giugno 2020 i termini di efficacia applicativa degli strumenti organizzativi previsti dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato e integrato. Tengo a rimarcare che, in ogni fase dell'emergenza, il Ministero ha fornito agli uffici giudiziari ogni forma di assistenza nell'organizzazione dell'attività giurisdizionale, anche attraverso circolari generali, volte a fornire indicazioni per garantire la tendenziale uniformità delle modalità di esercizio dei poteri organizzativi affidati espressamente dal legislatore ai dirigenti di ogni ufficio giudiziario. Ricordo, ad esempio, le circolari del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, datate 2 maggio 2020 e 12 giugno 2020, emanate proprio in vista della ripresa a pieno regime dell'attività giudiziaria. Fin dalla prima fase dell'emergenza è stata evidenziata la necessità di adottare misure organizzative e logistiche volte alla tutela della salute e dell'igiene degli ambienti e della sicurezza dei locali. Gli uffici giudiziari sono stati immediatamente autorizzati ad effettuare acquisti diretti di materiale igienico-sanitario, nonché un adeguato numero di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È stata, inoltre, prevista una procedura semplificata per la gestione delle richieste provenienti dagli uffici giudiziari, relative a pareti in plexiglass e a paratie parafiato è stata elaborata una serie di strumenti di controllo della temperatura. Si stanno inoltre offrendo supporto e indicazione agli uffici in merito alla pulizia e alla igienizzazione degli impianti di areazione nel periodo estivo. Corollario delle misure più spiccatamente a carattere igienico e sanitario rimangono quelle logistiche e organizzative, tra le quali: la regolamentazione dell'accesso ai servizi; l'istituzione di percorsi dedicati all'utenza; la gestione di una banca dati delle aule migliori, al fine di assicurare al meglio il distanziamento sociale e le altre prescrizioni sanitarie. Certamente, l'esigenza di mantenimento del distanziamento sociale si interseca con il problema degli spazi, soprattutto in ragione della necessità della ripresa delle attività giudiziarie cosiddette in presenza, con un aumento dell'afflusso dell'utenza, dei dipendenti, dei magistrati e degli avvocati, esigenza segnalata altresì dall'Ispettorato per la funzione pubblica, con note rivolte a vari uffici giudiziari. Sul punto, l'acquisizione di nuovi spazi a mezzo dell'utilizzo dello strumento di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 155 del 2012, che attribuisce al Ministero della giustizia la facoltà di accordarsi con Regioni e Province autonome per disporre temporaneamente l'utilizzo degli immobili delle cosiddette sedi giudiziarie soppresse, con retribuzione del personale e spese a carico del bilancio della Regione, non appare di immediata praticabilità, richiedendo tempi tecnici che non risultano compatibili con le esigenze di carattere emergenziale prospettate dagli interroganti. PRESIDENTE. sono stato abbastanza convincente, ma le assicuro che la mia richiesta è politicamente trasversale e corrisponde alle idee di tutti coloro che hanno a che fare con il mondo della giustizia, non soltanto nel tribunale cui ho fatto riferimento, Alba, in provincia di Cuneo, ma in tutta Italia, avendone parlato con colleghi di ogni partito. Lei sa che attorno ai tribunali chiusi e alle sedi soppresse si è verificata la desertificazione economica e sociale di intere zone, quartieri,

- salvo casi eccezionali - lo *smart working* nei tribunali, perché l'aula di un tribunale è un'altra cosa: è passione, è sensazioni, è una visione d'insieme, delle parti e delle richieste da parte dei giudici, del pubblico ministero, degli avvocati e degli imputati stessi. Nei fondi, di importo rilevante, a disposizione per il rilancio, forse c'è anche una piccola somma per la riapertura, che corrisponde all'economia reale e a funzioni giudiziarie

Gruppo Fratelli d'Italia sta cercando di trasferirle, senza risultati, tutta la preoccupazione per il momento che vive il mondo della scuola italiana. Abbiamo in ogni modo denunciato che il Governo aveva intrapreso strade sbagliate e scelte che hanno lasciato veramente molto perplesso - per usare un eufemismo - l'intero mondo della scuola.

completamente sbagliato, a nostro avviso) e non è stato accolto nessuno dei nostri suggerimenti, che riflettevano le richieste dell'intero mondo della scuola, dagli alunni alle famiglie, al personale docente e non docente, ai dirigenti scolastici. Non abbiamo neanche mancato, in quella sede, di rappresentarle tutta la preoccupazione

Apprendiamo dalle bozze dei decreti che svolazzano e dalle dichiarazioni, in un trionfo della formula del "salvo intese", che si ritiene di affidare al commissario Arcuri, che peraltro ha dato pessima prova di sé in occasione delle scelte legate all'emergenza Covid-19, le funzioni per il corretto avvio dell'anno scolastico. Le chiediamo in questa sede, che è la casa del popolo italiano, di cui noi siamo la rappresentanza, la conferma di questa decisione e le motivazioni per le quali il Ministero intende espropriarsi ed abdicare alle proprie responsabilità. Senatore Iannone, il Governo sta approntando tutte le misure affinché l'avvio del prossimo anno scolastico possa avvenire in modo ordinato e in piena sicurezza. L'articolo 235 del decreto-legge rilancio istituisce presso il Ministero dell'istruzione un fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, proprio per l'adozione degli interventi necessari alla riapertura delle istituzioni scolastiche e contenendo il rischio epidemiologico. Come preannunciato, a breve questo stanziamento sarà incrementato. Con tali risorse finanziarie si potrà derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe e attivare ulteriori posti di personale docente e ATA a tempo determinato per il prossimo anno scolastico. Per la prima volta dopo anni si potranno così ridurre le classi troppo affollate, anche grazie all'acquisizione di spazi supplementari sulla base delle necessità emergenti dei singoli territori, grazie al lavoro dei tavoli regionali appositamente costituiti. Inoltre, il menzionato decreto-legge ha incrementato il fondo per il funzionamento delle scuole di 331 milioni di euro per la pulizia e la costante igienizzazione degli ambienti scolastici, oltre che proprio per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Questi fondi sono già stati erogati alle istituzioni scolastiche e potranno essere spesi anche per piccoli interventi di manutenzione utili ad ampliare la disponibilità delle aule. La dirigenza scolastica non è stato affatto lasciata sola a fronteggiare i problemi. È forte l'impegno del Ministero, in tutte le sue componenti, anche periferiche, nell'affrontare insieme ai dirigenti scolastici, agli enti locali e agli altri attori istituzionali le criticità dei singoli territori e delle singole scuole, come sto direttamente sperimentando tramite la mia partecipazione ai singoli confronti regionali. È in questa ampia e articolata cornice di interventi posti in essere dal Governo che va collocata la proposta presente nel decreto-legge sulle semplificazioni di individuare il commissario per il coordinamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica quale soggetto che, in virtù dei poteri straordinari e derogatori, potrà acquistare e distribuire anche gli arredi scolastici. La scelta, già annunciata nel piano per la riapertura delle scuole varato lo scorso 26 giugno, di affidare questo compito precipuo ad una struttura commissariale già esistente è la più razionale: da un lato consentirà una maggiore tempestività negli acquisti, dall'altro eviterà diseconomie e duplicazioni. Colgo l'occasione, infine, per ringraziare il commissario Arcuri e la sua struttura che già si sta prodigando per far fronte a un nuovo, sfidante compito a favore della scuola pubblica del Paese.

Mi rendo conto che c'è un difetto di contatto con la realtà: evidentemente, lei non vede o non vuole vedere quello che la scuola italiana sta attraversando. Gli spazi non ci sono e si hanno difficoltà a reperirli; il personale, in questo momento, è impegnato a fare il geometra e, soprattutto, siamo ormai già alla metà di luglio. Lei dovrebbe sapere - chi ha fatto l'amministratore locale lo sa bene - che l'anno scolastico si programma con tempi ben diversi e, quindi, figuriamoci nella condizione post-emergenza che stiamo vivendo. Rimangono tutte le ansie, le angosce e i dubbi per gli alunni, le famiglie e il personale docente. Voglio ricordare quello che è stato fatto ai nostri insegnanti precari, ai diplomati magistrali che l'altro giorno manifestavano davanti alla sede del suo Ministero, ai precari di terza fascia che questa mattina erano a Montecitorio, tutti preoccupati per le tabelle per la valutazione dei titoli. preoccuparsi realmente della scuola italiana necessita anzitutto di uno sforzo di comprensione delle reali esigenze. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, affidarsi al commissario Arcuri, dopo quello che abbiamo visto durante l'emergenza - i ritardi e le discrasie delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale e tutte le mancanze del Governo nei confronti dei cittadini - equivale ad affidare la presidenza dell'Avis al conte Dracula.

da quanto si apprende da notizie di stampa il Governo, nel cosiddetto decreto semplificazioni, ha affidato al commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri la gestione della ripartenza dell'anno scolastico 2020-2021. Dopo aver esautorato il Parlamento delle sue funzioni, il Governo si appresta a fare lo stesso con i componenti dell'Esecutivo. Fino a oggi sono emerse tutte le criticità che hanno caratterizzato i provvedimenti governativi in materia scolastica emanati a seguito dell'emergenza Covid, a cominciare dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», nel quale molti aspetti inerenti la gestione della riapertura delle scuole in presenza a settembre non hanno trovato un'adeguata soluzione. Anche in fase di conversione sono rimaste molte incertezze, soprattutto riguardo la possibilità di realizzazione del giusto distanziamento tra gli studenti, del reperimento degli spazi e del reclutamento degli insegnanti necessari. Solo a fine giugno sono state emanate le linee guida per la riapertura delle scuole: un compendio di indicazioni generiche e prive del necessario approfondimento tecnico, senza azioni, metodiche e tempi certi, nonostante la stesura sia stata affidata a un comitato tecnico-scientifico specificatamente nominato. Il presidente dell'associazione presidi ha segnalato che c'è necessità di 40.000 classi aggiuntive per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza. In recenti dichiarazioni il Ministro in indirizzo ha avanzato l'ipotesi di utilizzare altri spazi per creare aule, ma si tratta di soluzioni di cui ancora non si conosce la praticabilità effettiva. Totalmente ignorato, tra l'altro, il contributo che possono fornire con i loro spazi le 12.564 scuole paritarie presenti su tutto il territorio nazionale.

genitori hanno manifestato e continuano a farlo. Nel resto d'Europa le scuole sono state gradualmente riaperte nel rispetto delle norme di sicurezza, assicurando il pieno rispetto al diritto all'istruzione. Da un sondaggio dell'Autorità per le comunicazioni risulta che 10 ragazzi su 100 sono rimasti completamente esclusi dal processo di apprendimento *online* e un ulteriore 20 per cento ha potuto frequentare i corsi soltanto in modo saltuario

Quanto premesso è volto a sapere quali siano le motivazioni che hanno portato l'Esecutivo alla decisione di affidare al commissario straordinario Domenico Arcuri la gestione della ripresa dell'anno scolastico 2020-2021.

Senatrice Alessandrini, il suo quesito mi induce a precisare preliminarmente l'esatta portata della disposizione contenuta nel decreto-legge sulle semplificazioni. Diversamente da quanto sostiene, il commissario straordinario non è affatto incaricato della gestione della ripresa del prossimo anno scolastico. Con la disposizione in esame, infatti, si prevede esclusivamente che il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponga sino al termine dello stato d'emergenza degli speciali poteri conferiti in relazione ai soli acquisti delle dotazioni strumentali eventualmente necessarie a contenere e contrastare l'emergenza nelle istituzioni scolastiche. L'avvio del prossimo anno scolastico - come ho precisato più volte - è invece accompagnato e sostenuto costantemente dal Ministero dell'istruzione. A fianco delle scuole vi sono di fatti una cabina di regia nazionale, con compiti di coordinamento, e tavoli regionali insediati presso gli uffici territoriali del Ministero, cui - come ho già detto - sto partecipando personalmente. Ci stiamo impegnando per fornire soluzioni concrete, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Le linee guida da lei richiamate, già diramate a tutte le scuole, sono il frutto di confronto e condivisione con gli attori del mondo della scuola, le Regioni, gli enti locali e le forze sociali: non sono affatto generiche, ma vanno proprio in questa direzione. Alla descritta attività - costante e capillare - di rilevazione dei bisogni, di sintesi e di ricerca di soluzioni, come più volte ricordato, si affianca la concreta azione del Governo, che ha stanziato le risorse finanziarie necessarie all'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico. Ciò permetterà di incrementare fino a 50.000 unità il personale docente e ATA per il prossimo anno scolastico, sulla base delle concrete esigenze che emergeranno dai territori. Continuiamo a investire anche nell'innovazione tecnologica, proprio per superare quel divario digitale da lei richiamato e garantire a tutti, ma proprio a tutti, il diritto allo studio. Ricordo che il Comitato nazionale per la banda ultralarga ha approvato un importante piano scuola, prevedendo la ridestinazione di 400 milioni a favore delle scuole per portare la banda ultralarga alla porta di ciascun edificio scolastico e garantire alle scuole per cinque anni la gratuità del canone di connettività. Aggiungo che recentemente sono stati destinati alle scuole secondarie di secondo grado statali ulteriori 29 milioni di euro per finanziare le *smart class*. Voglio concludere ribadendo con fermezza che nessuno studente sarà lasciato indietro. Il Governo sta lavorando ogni giorno per garantire l'effettività del diritto allo studio, unitamente alla libertà di scelta educativa delle famiglie.

ancora una volta riceviamo da lei risposte che delineano un quadro di misure totalmente insoddisfacente e la delusione non è solo la mia e del mio partito, Lega-Salvini Premier, ma è anche di tutto il mondo della scuola e di tutti i padri e le madri che che si aspettavano sicuramente ben altro da lei e dal Governo. Ministro, attualmente ho due certezze: la prima è che lei non sia in grado di gestire la scuola in una situazione di emergenza come questa *(Applausi)*; la seconda è che lei non sarebbe stata in grado di gestire la scuola nemmeno in una situazione di normalità. Se n'è accorto anche il suo *Premier*, che ha voluto commissariarla in alcune delle sue funzioni non ritenendola all'altezza di tale compito. Ministro, le chiedo, quindi, un atto d'amore nei confronti della scuola: si dimetta si dimetta dal suo incarico e lasci il suo posto a qualcuno di davvero competente.

il senatore Arrigoni, in quanto Questore, di aiutare aiutare la Presidenza e l'Assemblea a proseguire i lavori

signor Ministro, premesso che la scuola italiana ha saputo reagire alla crisi causata dal coronavirus con diverse misure eccezionali, tra le quali la didattica a distanza, gli insegnanti si sono attivati immediatamente provvedendo sia alla loro formazione, laddove mancava, sia a offrire, fin dove possibile, un adeguato servizio agli studenti. Tuttavia, non si può negare che la didattica a distanza abbia funzionato soltanto in parte: in alcune parti del Paese la linea Internet si è rivelata scarsa. Alcuni studenti sono rimasti sprovvisti degli strumenti informatici; per molti altri - mi riferisco, in particolare, agli alunni della scuola primaria e penso anche alla mia bambina di otto anni - la didattica a distanza non è mai partita, in quanto i compiti sono stati inviati mediante *mail* e WhatsApp per diversi mesi e poi su una piattaforma *on-line*, ma senza poter usufruire di alcuna video lezione in diretta *streaming*. La didattica a distanza ha caricato sul contesto familiare una serie di incombenze sia economiche che in termini di supporto e tempo che non tutti i genitori potevano permettersi, lavorando fuori casa e alcuni in *smart working*. Seppure utile nel breve periodo legato proprio alla gestione dell'emergenza sanitaria e nonostante gli ingenti stanziamenti del Governo, la didattica a distanza nel lungo periodo potrebbe determinare forti disuguaglianze, con danno soprattutto nei confronti dei soggetti più vulnerabili. La dispersione scolastica è già abbastanza alta in Italia e alla fine dell'emergenza potrebbe risultare più alta. Infine, poiché la scuola deve offrire non soltanto un piano didattico, ma anche un piano educativo e sociale e poiché, di conseguenza, appare necessario che a settembre 2020 tutti gli studenti, a partire dalle fasce dei più piccoli, possano rientrare in classe in una situazione di sicurezza, le chiedo quali strumenti il Governo stia mettendo in campo per consentire l'inizio armonioso e in sicurezza del nuovo anno scolastico 2020-2021.

alle nostre studentesse e ai nostri studenti, soprattutto quelli più in difficoltà e con svantaggio, che rischiavano di amplificare i divari territoriali e sociali già esistenti che abbiamo il dovere di ridurre e combattere. Per tale ragione, abbiamo investito da subito ingenti risorse per l'acquisto di *tablet*, di connessioni e di tutti gli strumenti digitali utili a vantaggio dei meno abbienti. Dall'inizio dell'emergenza, anche per sostenere la didattica a distanza, sono stati stanziati più di 180 milioni di euro; risorse che rimarranno alla scuola italiana, arricchendola. *Tablet* e *personal computer*, che abbiamo acquistato per sostenere i nostri ragazzi nella didattica a distanza, saranno adesso un patrimonio per il lavoro in classe e nei laboratori. La priorità di questo Esecutivo è stata e sarà sempre quella di non lasciare indietro nessuno. Anche per questo, nei giorni scorsi abbiamo varato un ulteriore avviso per complessivi 236 milioni di euro, a valere sui PON, che serviranno all'acquisto di libri *kit* didattici per oltre 750.000 nostri studenti e nostre studentesse più svantaggiati: una misura molto importante per il diritto allo studio e per la ripartenza a settembre che darà sostegno alle famiglie. Ogni scuola secondaria di primo grado potrà avere fino a 100.000 euro e le scuole secondarie di secondo grado fino a 120.000 euro. In questo contesto l'avvio del nuovo anno scolastico rappresenta sicuramente una sfida. Il Governo sta affrontando tutte le misure necessarie per la realizzazione di un ambizioso disegno: avere un organico potenziato, evitare classi sovraffollate, disporre degli spazi supplementari, laddove fossero necessari. La spesa per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ha registrato, in costanza dell'emergenza epidemiologica, un'accelerazione: a marzo scorso sono stati stanziati ben 510 milioni di euro; altri 320 milioni sono stati ripartiti tra le Regioni ad aprile; sono stati messi a disposizione ulteriori 855 milioni di euro a favore di Province e Città metropolitane. Inoltre, sono stati pubblicati i risultati relativi al bando che ha messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di azioni di cosiddetta edilizia leggera, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Nella concreta declinazione degli interventi da realizzare, le scuole non saranno lasciate sole. La stesura di uno specifico protocollo di sicurezza, sul modello di quanto già fatto per gli esami di stato, accompagnerà l'avvio del prossimo anno scolastico. Io stessa ho iniziato a partecipare ai tavoli tecnici regionali convocati per analizzare ogni situazione e trovare risposte adeguate insieme agli enti competenti - gli enti locali - in un'ottica di condivisione e celerità. A queste attività si affiancheranno già dalle prossime settimane appositi spazi di formazione per tutto il personale scolastico sulle tematiche digitali e sulla sicurezza. Posso rassicurarla che il Governo accompagnerà ogni passaggio del ritorno a scuola in presenza delle nostre studentesse e dei nostri studenti. *(Applausi).*

Signor Presidente, vorrei ringraziare il Ministro per aver risposto in maniera soddisfacente alla domanda postale.

Gelmini di 8 miliardi di euro. I signori che tirano fuori gli striscioni e dicono a lei di dimettersi sono quelli che hanno sostenuto le politiche di tagli alla scuola statale pubblica per 8 miliardi di euro. Lei, Ministro, è riuscita ad ottenere per la scuola statale pubblica 5,6 miliardi di euro, che saranno investiti per poter consentire il rientro in sicurezza dei nostri studenti e per migliorare lo stato di salute delle nostre istituzioni scolastiche. Ricordiamo che l'autonomia scolastica è stata un'iniziativa delle altre forze politiche che ci hanno governato in questi ultimi vent'anni, per cui adesso non possono certamente essere proprio loro ad attribuire a lei la responsabilità delle leggi con le quali si è ritrovata a dover operare, nel rispetto degli enti locali, delle autonomie scolastiche e, quindi, delle prerogative di tutti i soggetti che in questo momento sono chiamati a collaborare per risolvere l'emergenza in corso.

Comunico all'Assemblea che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare a conoscenza dell'Aula la situazione paradossale che si sta verificando in Umbria relativamente al potenziamento della rete ospedaliera per

con il Governo, alla fine la Regione ha ottenuto 50 posti aggiuntivi per un totale di 119 posti che permetteranno anche di soddisfare le esigenze di terapia intensiva degli eventuali malati Covid sia di chi, purtroppo, avrà eventualmente necessità di terapia intensiva per patologie non legate al Covid. tutto bene, perché il piano di riparto prevedeva che 42 posti andassero in tutte le strutture DEA di primo e secondo livello, che sono sette, e i nella struttura di Pantalla, che è stato il Covid Hospital regionale ad uso esclusivo. Peraltro, tutti i sindaci di qualsiasi colore politico hanno accettato questa decisione e hanno contribuito al potenziamento. Purtroppo il Governo ha rifiutato questo riparto perché

di subintensiva e quattro di intensiva. Servirebbe, quindi, semplicemente che le circolari dicano che, dove sono presenti realmente e fisicamente gli apparati, si possono

al Governo e l'appello affinché non si perda un'occasione e non si pieghi la realtà alla burocrazia, ma si pieghi la burocrazia al buon senso e si mantenga quello che già c'è e non costerebbe un euro in più e per il quale hanno contribuito anche gli enti locali e i privati.

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (1874).